per consentire - così si è espressa la Conferenza dei Capigruppo - ai senatori in missione a Strasburgo per i lavori della 14a Commissione sugli affari europei di essere presenti al momento del voto.

la mozione che mi accingo ad illustrare ha come argomento i rapporti tra il nostro Paese e la Libia. La Libia occupa una posizione di grande rilievo nel contesto nord-africano, anche per tutti i rapporti e i coinvolgimenti

devono essere continuamente rafforzati, con una capacità di reciproca collaborazione, finalizzata al miglioramento di tali rapporti e alla soluzione dei gravi problemi che attanagliano l'umanità ed in particolare quest'area del mondo. Si tratta di continuare a rafforzare quell'opera messa in atto soprattutto dall'allora ministro Pisanu, primo firmatario di questa mozione, e di chiudere, in via definitiva, quel contenzioso storico che, indubbiamente, ha caratterizzato

e che il Parlamento ha ratificato nel 2003. Si tratta di superare le esperienze negative del passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro della cooperazione tra i nostri due Paesi. dicevo, la collaborazione tra l'Italia e la Libia riveste importanza strategica per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo, come pure per il conseguimento del dialogo euro-africano. Tutto ciò - lo sottolineo con forza e determinazione perché è l'elemento che deve caratterizzare il rafforzamento di questo rapporto - deve avvenire in un ambito sempre più stretto fra l'Europa e il Nord-Africa. In tal senso, l'Italia ha svolto - come dirò in seguito - un ruolo veramente fondamentale per raccordare meglio, con reciproca soddisfazione, i rapporti tra l'Europa, la Libia e il Nord-Africa. Nord-Africa. In occasione del dibattito parlamentare che si svolse il 22 febbraio 2006 di fronte alle Commissioni affari costituzionali e affari esteri riunite del Senato e della Camera, il Governo, con gli allora ministri Fini e Pisanu, confermò l'impegno a proseguire l'intensa azione svolta e ad adottare tutte le possibili iniziative per dare impulso e vigore al partenariato tra l'Italia e la Libia, anche sulla base di una fruttuosa cooperazione in atto contro la lotta all'immigrazione clandestina e le operazioni criminali. Si sono così messe in pratica azioni concrete necessarie a chiudere il capitolo storico del passato coloniale, nonché le ulteriori fasi altamente significative di cooperazione privilegiata, concordate sempre con la parte libica, che hanno confermato il segno dell'amicizia e della collaborazione tra i due Governi e i due popoli. Contemporaneamente, era anche necessario che le autorità libiche dessero seguito concreto agli impegni sottoscritti, in particolar modo ai fini della concessione, senza limitazione e discriminazioni, dei visti ai profughi italiani. Era altresì necessario ricercare, sempre d'intesa con la parte libica, una accettabile ed equa soluzione del contenzioso economico sui crediti che le aziende italiane vantavano, in modo anche da superare le discriminazioni sul piano normativo a danno delle imprese italiane operanti in Libia. Questi impegni furono definiti a seguito del dibattito successivo ai gravi episodi che si svolsero a Bengasi nel febbraio 2006. In quella tragica occasione (lo ricordo, e lo voglio sottolineare, perché quando esistono rapporti estremamente amichevoli, di comprensione e di capacità di comprendere i problemi, questi vengono risolti con più facilità), ci fu una lunga ed amichevole conversazione telefonica tra il presidente del Consiglio Berlusconi, e il *leader* Gheddafi: quest'ultimo espresse rammarico per gli episodi di Bengasi il presidente Berlusconi espresse profondo dolore per le vittime, ringraziando per gli interventi delle forze di polizia che avevano consentito di portare in luogo sicuro il personale italiano, confermando che il grave episodio non doveva ripercuotersi negativamente sui rapporti fra i due Paesi e anche sul loro ulteriore sviluppo. Si osservò che quell'ondata di violenza scatenata dall'integralismo islamista aveva come vittime innanzi tutto la stragrande maggioranza silenziosa di credenti di fede islamica. Dunque, era proprio quest'ultima che poteva opporsi alla violenza dei fondamentalisti. Si affermò che l'unica strada per rafforzare questa maggioranza e l'autorevolezza dei Governi moderati è quella del dialogo costruttivo, responsabile e svolto con tanta pazienza, ma anche con tanta determinazione. Da qui il dialogo, la cooperazione e il rafforzamento delle relazioni bilaterali, realizzate anche con frequenti missioni del Governo, con tutti i Paesi dell'area e quindi in particolare anche con la Libia. L'azione dell'Italia è avvenuta naturalmente in ambito europeo, come sottolineavo: da qui anche l'impegno per la revoca delle misure restrittive adottate nei confronti della Libia, avvenuta in data 14 ottobre 2004, e successivamente nella consapevolezza che il problema delle migrazioni potesse essere affrontato con più efficacia nell'ambito di una più stretta collaborazione tra Unione Europea e Paesi africani. L'Italia si è impegnata a far sì che L'Unione Europea avviasse una specifica collaborazione con la Libia e il Consiglio Europeo del dicembre 2005 ha confermato il carattere prioritario dei programmi euro-libici nel contesto di un approccio globale euro-africano relativo al problema delle migrazioni. Sia la Commissione che il Parlamento europeo hanno riconosciuto la collaborazione bilaterale italo-libica come valido modello su cui basare le iniziative comunitarie. Del resto, c'è una convergenza di problemi per la cui soluzione è fondamentale una stretta, reciproca collaborazione. La Libia è un Paese esposto a intense migrazioni illegali e ai conseguenti fenomeni criminali, soprattutto per l'instabilità politica del Corno d'Africa per le terribili carestie della fascia subsahariana che inducono una forte pressione alle sue frontiere desertiche. Io qui ricordo quello che da troppo tempo sta avvenendo in tante zone dell'Africa dove, purtroppo, ci sono ancora situazioni che non possono che essere denominate come genocidi, e penso al Darfur. Ecco qual è il grande problema, ecco dove sta la grande sfida dei rapporti tra l'Europa e questo grande continente, per il quale dobbiamo lavorare assiduamente e dobbiamo creare tutte le condizioni per affrontare concretamente tali problemi, perché se non si riesce a farlo (e io qui dirò quali elementi sono alla base di questo rapporto), se non c'è concretezza operativa, è chiaro che le parole sono dette al vento e non si riesce, appunto, a risolvere questi immensi problemi del pianeta. La Libia, dicevo, in relazione a questo contesto geopolitico, è diventata il Paese verso il quale si convoglia gran parte dell'emigrazione clandestina,

problema della tratta degli esseri umani. È un problema veramente scandaloso nei confronti del quale dobbiamo mettere in atto tutte quelle misure e quelle capacità per debellare quella che è la nuova schiavitù di questo secolo, quella che è la grande piaga di questa nostra epoca. Sono stati di grande rilievo i risultati ottenuti dalla collaborazione tra le forze di polizia di Libia e Italia in contrasto verso questo fenomeno, la tratta degli esseri umani e la trasmigrazione, che costantemente In occasione della citata seduta del 22 febbraio 2006, il ministro Pisanu riferiva i dati forniti dal Governo di Tripoli: oltre 44.000 clandestini bloccati prima della partenza per l'Italia, 5.500 persone arrestate per reati connessi all'immigrazione clandestina, 45 associazioni criminali sgominate *in loco*. Grazie alla collaborazione delle autorità libiche, in Italia, in quel periodo, sono state arrestate 2.800 persone e denunciate altre 7.000. Risultati, questi, in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di droga e all'immigrazione clandestina, che trovano origine nella cooperazione italo-libica in base ad un accordo ratificato dal Parlamento nel 2003. In relazione all'immigrazione clandestina, l'accordo prevedeva la reciproca assistenza, lo scambio di informazioni sui flussi migratori e sulle organizzazioni criminali che li gestiscono e li sfruttano anche atrocemente. Ricordo che nell'estate del 2003, sulla base dello stesso accordo, il ministro dell'interno Pisanu aveva raggiunto ulteriori intese operative con l'omologo Ministro libico per rafforzare la lotta ai trafficanti di esseri umani e avviare così un programma articolato di assistenza tecnica. Sempre in base a quell'accordo, vi è stata una notevole attività di formazione professionale, in particolare a favore di 500 ufficiali della polizia libica. Vi è stato il rimpatrio verso i Paesi terzi di clandestini diretti in Italia e rintracciati dalle autorità libiche. Una consistente fornitura di mezzi ed equipaggiamenti tecnici dedicati al soccorso e all'assistenza dei clandestini. Un impegno veramente consistente e notevole in rapporto a tale riguardo con la Libia, se si pensa che l'impegno economico in tal senso ha rappresentato circa il 50 per cento delle risorse messe a disposizione dalla Direzione centrale dell'emigrazione e della Polizia centrale delle frontiere. frontiere. E ancora, realizzazione di centri per immigrati clandestini, destinatari di provvedimenti di allontanamento dal territorio libico. Collaborazione operativa ed investigativa con esperti italiani distaccati presso l'ambasciata italiana a Tripoli, anche con l'obiettivo di costruire squadre investigative miste. E ancora, sviluppo della cooperazione regionale e della capacità istituzionale della Libia e del Niger nel campo della gestione delle frontiere e del contrasto all'immigrazione clandestina: il progetto, denominato «*Across Sahara*», è cofinanziato dalla Commissione europea all'80 per cento, pari ad un importo di 1,5 milioni di euro. Per l'implementazione del progetto è prevista anche la fornitura alla Libia e al Niger di alcuni veicoli fuoristrada e di tutta una serie di attrezzature. In attuazione degli accordi di collaborazione con la Libia per il contrasto all'immigrazione vi è stata poi una delegazione di esperti italiani che si è recata a Tripoli per effettuare un'approfondita analisi dell'attuale capacità operativa della polizia libica. Al termine della missione, è stato redatto un progetto per la creazione in Libia di un apparato di polizia di frontiera terrestre e marittima, comprensivo anche della fornitura di armamenti, equipaggiamenti, con una previsione di spesa consistente di 7 milioni di euro, nonché progetti di formazione - questo è il punto centrale e fondamentale - per altri 5 milioni di euro. E poi ci sono stati incontri con esperti di alto livello in Italia, a Malta, in Libia, della Commissione europea incaricati di elaborare proposte per rafforzare la collaborazione tra l'Unione Europea e la Libia in materia di contrasto all'immigrazione illegale. Tutti questi sono elementi concreti; sono tutte forme di collaborazione che hanno rinsaldato i rapporti fondamentali, direi strategici, tra l'Italia e la Libia, nel più ampio dialogo euro-africano. Risultati poi di questa collaborazione e del rafforzamento dei rapporti amichevoli con la Libia sono stati anche il ritorno di alcune nostre grandi aziende (cito ENI, la Finmeccanica) che hanno consentito di rafforzare le relazioni economiche e quindi anche strategiche tra i nostri due Paesi. La Libia, dunque, come Paese amico, un *partner* determinato nella lotta al terrorismo e alle organizzazioni criminali che mettono in atto traffici di esseri umani e di droga; traffici che devono essere debellati con la massima determinazione. C'è anche il contesto - cui ho fatto cenno all'inizio - dell'integralismo e del terrorismo. Da qui la necessità di discutere e operare proficuamente con l'Islam moderato, sia quello largamente maggioritario nelle comunità musulmane in Europa, sia quello dei Governi laici della sponda meridionale del Mediterraneo e del Medioriente. sono le grandi sfide e i rapporti sviluppati proficuamente tra l'Italia e la Libia in tutto questo contesto per il conseguimento di obiettivi fondamentali per la pace e lo sviluppo possono e devono essere continuati e rafforzati ulteriormente. Il ministro dell'interno, onorevole Pisanu, nel concludere i lavori della citata seduta congiunta del 22 febbraio 2006, che vide un grande consenso su questi temi,

«un'esortazione a procedere sulla via della collaborazione con il mondo islamico e a intensificare i rapporti con la Libia che è, per tanti aspetti, Paese cruciale nelle relazioni mediterranee» e anche del dialogo euro-africano. È questo, in sintesi, l'impegno che si chiede al Governo con la mozione n. 48. Il Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2006 come citato nella mozione - aveva deliberato di «adottare tutte le iniziative opportune a dare respiro strategico e forte valenza operativa alla *partnership* Italia-Libia»; Governo a favorire, con il potenziamento dei rapporti bilaterali Italia-Libia, anche il dialogo euro-africano e la cooperazione fondamentale nell'area mediterranea. È quanto si chiede al Governo per continuare l'opera difficile, ma determinata e con positivi risultati sviluppata dal precedente Governo. Mi auguro, signor Presidente, che vi sia un ampio consenso in quest'Aula per fare in modo che tale attività, sviluppata con impegno e con tanta intensità, possa ottenere risultati positivi, perché ne va dell'equilibrio e della capacità di rafforzare la grande area del Mediterraneo.

per impegnare il Governo - e non perché oggi il Governo non sia impegnato - a portare avanti relazioni sempre più proficue con la Libia, ma perché rimangono problemi aperti che il Parlamento ha il dovere di sottolineare per ricercarne al più presto una soluzione. I rapporti con la Libia hanno conosciuto fasi alterne nel corso degli anni in particolare in tutto il periodo del dopoguerra. Un passo avanti per normalizzare le relazioni a livello politico e dei Governi è stato fatto nel 1998, quando fu firmato un comunicato congiunto congiunto inteso a porre fine alle *querelle* del passato, quelle che i libici hanno considerato le sofferenze del periodo coloniale, e a stabilire rapporti su una nuova base. In effetti, quel comunicato è stato la base delle relazioni fra i nostri due Paesi da quel momento in poi. Infatti, anche se con fasi alterne, perché episodi negativi vi sono stati, il rapporto fra i nostri due Paesi si è continuamente rafforzato. Già nel 1998 i due Governi esprimevano la loro volontà e determinazione a sviluppare relazioni bilaterali su nuove basi fondate sull'uguaglianza, il mutuo rispetto e la reciproca collaborazione nei vari campi, per promuovere gli interessi e il benessere dei nostri popoli e contribuire al sostegno della pace e della stabilità nella regione del Mediterraneo, al suo sviluppo economico e al benessere dei suoi popoli. Quel comunicato intese risolvere una serie di problemi, in particolare il problema della riammissione in Libia degli italiani espulsi, non soltanto per ragioni di visita o di turismo, ma anche di lavoro. posero le basi per la soluzione dei crediti rimasti in sospeso fra i nostri due Paesi. ha riconosciuto la validità di un gran numero di progetti e di contratti, ma ne rimangono ancora in sospeso. Quindi è bene cercare di ottenere la parte rimanente di quei crediti, sottolineando al Governo l'importanza di questo aspetto. Un'altra questione importante trattata nel comunicato congiunto del 1998 riguardava i problemi dello sminamento del territorio libico. A tale riguardo l'Italia ha dato un contributo fattivo. Inoltre ha ha finanziato la costruzione di un ospedale per le protesi per coloro che venissero colpiti o feriti dalle mine che ancora si trovano sul territorio libico,

Purtroppo, ogni tanto succede ancora che qualcuno cammini per quel deserto e venga colpito da mine. Una grande sensibilità a tale riguardo è sempre stata espressa dal Governo libico. Inoltre, già a quell'epoca l'Italia ha dato, attraverso il comunicato congiunto, un grande contributo nel campo culturale e sanitario, ammettendo studenti libici nelle nostre università, accettando nelle nostre strutture sanitarie malati libici che non possono trovare adeguata adeguata assistenza sul territorio libico, e in altri settori, come quello della restituzione delle opere d'arte trafugate. A quell'epoca, anche con la costituzione di una società mista italo-libica, si erano poste le condizioni per rapporti solidi fra i nostri due Paesi. Questi rapporti si sono sviluppati - dicevo - con fasi alterne: vi è stato l'episodio di Bengasi**,** di cui il Parlamento si è occupato (in particolare nell'audizione congiunta del 22 febbraio 2006). I rapporti però, nonostante questi episodi, sono sempre rimasti improntati ad amicizia e collaborazione. L'Italia è il principale *partner* economico della Libia. Per noi questo è di grande rilievo, non solo per i grandi investimenti effettuati nel campo dell'esplorazione e quindi nel campo energetico, petrolifero e del gas,

Lo sforzo di contrasto all'immigrazione clandestina da parte libica subisce rallentamenti quando vi sono questioni politiche aperte fra i nostri due Paesi che non trovano soluzione. Credo che sia il Governo di centro-sinistra fino al 2001 che quello di centro-destra negli anni successivi fino al 2006, si siano fortemente impegnati affinché si potesse ottenere una collaborazione piena da parte della Libia nella lotta all'immigrazione clandestina. Da parte libica si nota

indipendentemente dalla volontà delle autorità libiche di controllo dell'immigrazione clandestina spesso

al dialogo euro-africano. La Libia è parte del processo di Barcellona e anche del Gruppo dei cinque più cinque, al quale la Libia attribuisce grande importanza. Si tratta, cinque Paesi della sponda nord e di cinque Paesi della sponda sud del Mediterraneo, nel quale si confrontano opinioni e si cerca di rafforzare la collaborazione, in particolare fra i nostri Paesi europei e i libici. Credo sia importante proseguire il dialogo e rafforzare il rapporto di amicizia fra i nostri due Paesi. Per l'Italia credo che la Libia sia un *partner* strategico e che, nonostante le difficoltà che a volte emergono, sia importante proseguire dialogare con il Governo libico, un Governo non facile in ogni momento, ma con il quale credo dobbiamo assolutamente impegnarci per rafforzare la collaborazione. Rimangono alcune questioni aperte che queste mozioni intendono portare all'attenzione del Governo, in particolare la necessità fine al passato coloniale con opere e azioni che rappresentino in modo significativo la volontà del nostro Paese di porre fine a un capitolo della storia italiana e libica. La Libia si attende un grande gesto da parte dell'Italia, che possa essere visto e riconosciuto come un gesto di grande amicizia del nostro Paese nei suoi riguardi e questo e questo dovrebbe concretizzarsi con un'opera infrastrutturale. Credo che ci sia l'impegno di ricercare le risorse necessarie un'infrastruttura stradale importante - una strada o anche il suo progetto - che porti il nome dell'Italia, per mostrare l'amicizia del popolo italiano

poi la questione relativa ai crediti e credo che anche questa possa essere di nuovo affrontata. Non è che la Libia sia un Paese povero. Ritengo vi sia la volontà di risolvere tali questioni pendenti, di crediti, di contratti non riconosciuti o non andati a buon fine (il contenzioso nasce da ciò, non dalla mancanza della volontà libica di

relazione fatta dal collega Pianetta e credo che vi sia la volontà, certamente da parte nostra, della maggioranza - ma mi pare anche dell'opposizione di addivenire all'approvazione da parte del Senato di una mozione che impegni maggiormente il Governo alla soluzione delle questioni che rimangono ancora aperte, nell'interesse reciproco, sia della Libia sia dell'Italia. Quindi, mi auguro che la discussione che seguirà possa portare a un vasto consenso sul contenuto del documento al

*(UDC)*. Signor Presidente, le relazioni tra l'Italia e la Libia sono uno dei punti centrali della nostra politica estera e non da oggi, direi almeno dall'inizio di questo secolo: relazioni difficili che sono entrate profondamente anche nell'autodefinizione della coscienza nazionale, sia del popolo libico sia del popolo italiano. Siamo andati in Libia nel 1911 con una breve guerra, a cui è seguito un lungo periodo di occupazione e di guerriglia. In Libia nasce, almeno in parte, il mito dell'italiano «brava gente»: un modello di colonialismo diverso da quello di altri Paesi, capace di portare le strade, le scuole e di stabilire rapporti positivi con la popolazione locale. Ma - ahimè - questa è soltanto una metà della nostra presenza in Libia; c'è un'altra metà, quella della repressione, delle deportazioni di popolazioni innocenti, delle esecuzioni sommarie, che ci mette, non - come ha detto qualcuno - sullo stesso piano dei nazionalsocialisti, ma certamente su un piano non molto diverso da altre potenze coloniali (come la Francia in Algeria, la Gran Bretagna in Kenya e in altri Paesi) e che ha lasciato un durevole strascico. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, re Idris scelse consapevolmente di puntare sull'aspetto positivo della collaborazione italo-libica. All'inizio del Governo di Gheddafi, dopo il rivolgimento che lo portò al potere, vi fu una svolta, un diverso modo di pensare la memoria storica e, di conseguenza, un diverso rapporto con l'Italia. Avvenne il recupero degli eroi della resistenza antitaliana

si è tentato. In questo ambito, il Governo Berlusconi, talvolta demonizzato come contrario al multilateralismo e servo degli americani, ha adottato iniziative in perfetta continuità con una politica estera direi «andreottiana» e, con notevole indipendenza anche rispetto agli Stati Uniti, è stato il precursore dell'apertura di un rapporto nuovo con la Libia. Sapete del coinvolgimento affermato del regime di Gheddafi con atti di terrorismo e delle rappresaglie a cui ciò ha portato; tutto questo processo segna un passaggio improvviso con l'affermarsi dell'integralismo islamico. La dottrina sulla base della quale Gheddafi tenta di organizzare il proprio il proprio Stato - anche se i libici contestano la traduzione di Jamahiriya con la parola Stato - è fondamentalmente laica, fa riferimento a diritti umani universali e si trova spiazzata dall'emergere del radicalismo islamico che le si oppone con grande decisione e energia e al quale anch'essa si oppone con pari decisione e energia. Questo genera anche un cambiamento di politica estera e una maggiore disponibilità a parlare con l'Occidente, in cui si inseriscono le iniziative diplomatiche italiane, dal

proprio il nuovo atteggiamento del Governo Gheddafi, insieme a quello del Governo Mubarak in Egitto, un pilastro dell'Occidente in generale, ci permette di separare le problematiche del Mediterraneo occidentale,

che rischiano di trovarsi in una missione impossibile: vanno in Libano per aiutare il Governo libanese a disarmare *Hezbollah,* che non vuole essere disarmato e che il Governo libanese non è in grado di disarmare. Dovremo pur fare, un giorno, una riflessione

del Mediterraneo occidentale, un'area relativamente più pacifica in cui il terrorismo è sotto controllo, anche dopo l'avviarsi a conclusione della guerra civile in Algeria,

È necessaria una politica integrata europea che contempli campi di accoglienza in territorio libico, cosa che consente di offrire un aiuto umanitario e anche di controllare questi movimenti di popolazione; è necessaria una politica europea per l'acqua a Sud del Sahara,

e, notando la convergenza delle due mozioni presentate, credo che forse sarebbe opportuno fare uno sforzo per unificarle e per dare ad esse una maggiore dimensione europea.

Solo attraverso la collaborazione degli Stati rivieraschi del Mediterraneo, infatti, possiamo contenere l'immigrazione clandestina. Abbiamo bisogno, contemporaneamente, di un'iniziativa europea a Sud del Sahara,

come anche quello di Lisbona: pare che in Europa, ogni qual volta dobbiamo coprire un'incapacità di agire, ci inventiamo un processo che però non cammina. Allora, il processo di Barcellona è sostanzialmente un fallimento, con una eccezione parziale per il Marocco. Bisogna farlo ripartire, realizzando un mercato comune del Mediterraneo meridionale. Oggi, tra la Libia,

Voglio ricordare, in questa occasione, una grande amica personale e dell'Italia, la signora Loyola De Palacio, recentemente scomparsa, che aveva lanciato l'idea dell'infrastrutturazione del lato meridionale del Mediterraneo, all'interno della quale si inserisce anche la domanda da parte della Libia di un forte sostegno italiano per costruire una grande linea di comunicazione, che vada da Bengasi a Torino. L'idea non è sbagliata, è sbagliato pensare che la finanzi l'Italia da sola, ma soprattutto è sbagliato pensare che questa infrastruttura possa essere isolata da una grande arteria che vada da Marrakesh fino al Cairo.

scisso dal recupero del Sud Sahara e dallo sviluppo economico del Maghreb, in una prospettiva europea. Non dobbiamo tacere, in questa occasione, una questione fondamentale, quella dell'evoluzione democratica del regime libico, del rispetto dei diritti umani.

Paesi, per le condizioni in cui si trovano, aperture improvvise potrebbero portare ad una prevalenza di movimenti islamici nostri nemici, come è successo in una certa fase in Algeria, ma sappiamo anche che non possiamo durevolmente, contro i nostri principi, mettere fra parentesi la questione della libertà. Vorrei suggerire di fare uno sforzo comune per mettere insieme, da un lato, il tema dei risarcimenti, affrontato nelle proposte di legge che ho ricordato, e dall'altro il tema della lotta all'immigrazione, collegato con quello dello sviluppo economico e della

i problemi sollevati. Oggi l'Europa non è molto popolare e tuttavia è soltanto a livello dell'Europa che si possono affrontare le grandi questioni della pace e della libertà. Dovrebbe essere una spinta per noi a a riprendere in mano, come propone ultimamente il cancelliere Angela Merkel, anche il disegno di un rafforzamento dell'Europa e della ripresa del processo costituzionale.

il Governo, guidato dall'allora presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, adottava una serie di decisioni volte a promuovere tutte le iniziative opportune per dare respiro strategico e forte valenza operativa alla *partnership* Italia-Libia, assegnando priorità assoluta alla duplice esigenza (che oggi ho visto richiamata saggiamente in diversi interventi in discussione generale)

e di continuare a ricercare, con la parte libica, una soluzione accettabile del contenzioso economico sui crediti che vantano le aziende italiane. Credo che, in questo contesto, ci sia una chiara continuità nelle scelte di politica estera. Lo ricordava il presidente Dini; gli atti

operando. Oggi abbiamo il problema di individuare un percorso per la risoluzione di questo insieme di contenziosi Italia-Libia e per il rilancio del dialogo bilaterale. Condivido molte delle riflessioni del senatore Buttiglione: il tema del rilancio delle relazioni bilaterali è strategico per l'Italia e per l'Unione Europea. Molte cose potranno essere affrontate soltanto in un rilancio strutturale dei rapporti strategici tra Unione Europea e Libia. In questo contesto, a partire dalla primavera del 2006, si sono moltiplicati i contatti al più alto livello tra il nuovo Governo italiano e le autorità libiche, che hanno finalmente portato alla nomina di un nuovo ambasciatore libico presso il Quirinale. L'ambasciatore Al Obeidi aveva, infatti, lasciato l'incarico nel 2004 e per quasi due anni non era stato più presentato un ambasciatore libico presso il Quirinale. Il 4 luglio ed il 3 agosto 2006, il vice presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, onorevole D'Alema, ha incontrato l'ambasciatore Al Obeidi. Tali incontri hanno confermato l'impegno di entrambe le parti a rilanciare il dialogo politico, per superare i contenziosi del passato e consentire il pieno sviluppo delle relazioni bilaterali in tutti i settori di mutuo interesse. Questi primi colloqui, dopo l'entrata in carica del nuovo Governo Prodi, hanno consentito di tracciare un percorso per il raggiungimento di un'intesa globale, che consenta la definitiva chiusura del capitolo del passato e di tutti i contenziosi bilaterali e ponga le basi per l'avvio di un forte partenariato di valenza strategica tra Italia e Libia. In tale contesto, la positiva soluzione della questione dei visti per gli esuli italiani dalla Libia e il ripagamento dei crediti dovuti da enti libici ad oltre un centinaio di imprese italiane assumono, ovviamente, un carattere prioritario nell'azione dei prossimi mesi. I successivi incontri avuti dal ministro D'Alema con il ministro degli esteri libico Shalgam nel settembre 2006 (a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York) e il successivo 14 dicembre a Roma hanno consentito di effettuare ulteriori passi in avanti per definire questa intesa bilaterale fortemente auspicata.

come il nostro obiettivo, peraltro condiviso con l'Esecutivo precedente, sia quello di porre le basi per uno sviluppo, su basi certe e concordate, di una *partnership* strategica tra i due Paesi, che quindi consenta di superare definitivamente il capitolo del passato e di favorire un pieno sviluppo dei rapporti in tutti i settori. Quando penso al raggiungimento di un'intesa globale, penso ovviamente alla alla risoluzione dei principali contenziosi che ancora creano un*vulnus* nei nostri rapporti: i visti per gli esuli italiani dalla Libia e il ripagamento dei crediti dovuti da diversi enti libici ad oltre cento imprese italiane. In questo contesto, penso che anche un dialogo strutturato sul tema dei diritti umani abbia un senso e una forza. Certo, si tratta di un Paese sovrano, ma l'Unione Europea ha attivato diversi luoghi di confronto sul tema dei diritti umani e sullo sviluppo del processo democratico. Ritengo che sia anche nell'interesse strategico della Libia compiere significativi passi in avanti ed è nostro interesse costruire *partnership* solide in grado, come una vera *partnership* strategica, anche di confrontare e di discutere i nodi critici. La Libia è sicuramente un Paese che può ancora compiere progressi nel settore della libertà religiosa e nel settore dei diritti fondamentali ed è nel nostro interesse esercitare una forma di positiva pressione, anche in un contesto di relazioni amichevoli, per favorire uno sviluppo sostanziale delle libertà e dei diritti fondamentali. Per quel che riguarda poi le relazioni tra l'Unione Europea e la Libia, vorrei sottolineare che il dialogo politico sulle tematiche dei rapporti euro-africani e della collaborazione nel Mediterraneo rappresentano una priorità, tanto per il Governo italiano quanto per quello libico. Tale priorità ha visto, nel comune impegno, la realizzazione della Conferenza Unione Europea-Africa sull'emigrazione e lo sviluppo, che si è svolta a Tripoli il 22-23 novembre del 2006. L'Italia guarda, inoltre, con favore al progressivo sviluppo dei rapporti fra Tripoli e l'Unione Europea non solo riguardo ai temi prioritari di collaborazione (penso alla lotta all'immigrazione clandestina), ma anche nell'ottica di una condivisione di quei valori che si auspica possano costituire un comune denominatore dell'area euro-mediterranea. In tale contesto, da parte italiana si rinnova anche l'auspicio - e l'abbiamo rinnovato in più di un'occasione - che la vicenda del personale sanitario bulgaro e palestinese, condannato a morte dalle corti libiche, possa trovare a breve una soluzione positiva. Si tratta di un caso nel quale,

il Governo condivide le istanze alla base delle due mozioni, sia quella presentata dal senatore Pisanu e illustrata dal senatore Pianetta, sia quella presentata dalla senatrice Finocchiaro e illustrata dal senatore Dini. Entrambe permettono di lavorare in un segno di forte continuità della politica estera in questo settore e attribuiscono, come attribuisce il Governo, un elevato grado di priorità al rilancio delle relazioni bilaterali Italia-Libia,

sul quale costruire una politica del nostro Paese in grado di chiudere definitivamente i contenziosi del passato e di aprire una stagione nuova che, inevitabilmente, sarà una stagione di sviluppo, anche di

del nostro Paese. Il Governo esprime pertanto parere favorevole su entrambi le mozioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto di questo pomeriggio potrà davvero segnare un punto di svolta storico nei rapporti italo-libici. Dal secondo dopoguerra ad oggi, tali rapporti hanno avuto un'evoluzione tormentata, ma non hanno mai registrato rotture insanabili, neppure nei momenti più difficili dello scontro con l'Occidente, dell'isolamento e della messa al bando della Libia nella comunità internazionale. Nonostante tutto, come sottolineò l'anno scorso in un dibattito qui al Senato il senatore Andreotti, Italia e Libia hanno saputo mantenere la necessaria concordia e consolidare proficui rapporti. Certamente ha pesato e continua a pesare come un macigno la memoria degli anni sanguinosi della prima e della seconda colonizzazione italiana; anni nei quali il popolo libico difese la sua dignità e conquistò la sua identità nazionale a prezzo di enormi sofferenze. Quel ricordo doloroso deve ora essere rimosso una volta per sempre. Certamente sono andate in questa direzione molte delle iniziative finora sostenute da entrambe le parti, ma non sono bastate.

e le successive intese operative stabilite dal Governo Berlusconi in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di esseri umani e all'immigrazione clandestina. Sulla scia di quelle intese, tra il 2003 e il 2004, l'Italia si è impegnata a fondo per la rimozione dell'embargo e per favorire, in ogni possibile modo, il reinserimento della Libia nella comunità internazionale. Un reinserimento per tanti aspetti meritato; non dimentichiamoci che alla vigilia dell'11 settembre il colonnello Gheddafi fu il primo *leader* arabo a denunciare l'estrema pericolosità di Al Qaeda e di Bin Laden e a suggerire una vasta iniziativa internazionale contro l'estremismo islamico impostata sul dialogo pacifico e il confronto delle culture. Allo stesso tempo, le autorità libiche avevano sottoscritto onerosi accordi per sistemare le tragiche partite di Lockerbie, Berlino e Uta e avevano dichiarato la rinuncia alle armi di distruzione di massa, aprendosi alla collaborazione internazionale per lo smantellamento del loro arsenale chimico. Ricordiamoci, inoltre, i dati poc'anzi illustrati dal collega Pianetta, che dimostrano con quale impegno la Libia, divenuta ormai principale Paese di transito dei grandi flussi migratori provenienti dal Continente africano e dal vicino Oriente, abbia collaborato con noi per contrastare l'immigrazione clandestina e combattere le organizzazioni criminali che la sfruttano spietatamente. Pur svolgendosi tra enormi difficoltà operative, quella collaborazione ha raccolto larghi apprezzamenti in Europa, come del resto ha confermato il successo della grande Conferenza internazionale conclusa a Tripoli il 23 novembre scorso con una importante dichiarazione congiunta tra Africa e Europa sui problemi delle migrazioni e dello sviluppo. Questi e numerosi altri fatti ci dicono, onorevoli senatori, che la Jamahiriya libica ha voltato pagina rispetto agli aggressivi anni Ottanta, contrassegnati dalle guerre lampo con l'Egitto e il Ciad, dagli scontri con gli americani e dal missile a Lampedusa. Oggi, mentre si accredita sul piano internazionale, la Libia rivede la sua organizzazione economica, sociale e istituzionale, cerca una propria, autonoma via alla modernità e si interroga su come la sponda Sud-occidentale del Mediterraneo possa collaborare con l'Europa per governare le migrazioni e porre argine al collasso economico e demografico del Continente africano. In questa prospettiva, l'Italia è percepita come un *partner* naturalmente privilegiato, sia per le sue buone relazioni politiche e culturali, che ho appena richiamato, sia per la ragguardevole e crescente cooperazione economica in numerosi campi di attività, non soltanto quello dell'energia. Ma perché questa *partnership* possa dispiegare tutte le sue potenzialità, occorre prima sistemare il complesso contenzioso ancora in discussione tra i due Paesi. Mi riferisco, in particolare, ai crediti vantati da diverse aziende italiane nei confronti della parte libica, agli ostacoli persistenti nella concessione dei visti di ingresso ai profughi italiani e, infine, al mancato accordo sul cosiddetto grande gesto che l'Italia deve compiere per chiudere definitivamente il capitolo storico del colonialismo. Proprio per questo, il 23 febbraio 2006, il Consiglio dei ministri, portando a conclusione un lungo confronto che aveva personalmente impegnato il *leader* libico Gheddafi e il presidente Berlusconi, deliberava di adottare tutte le iniziative necessarie per superare quel contenzioso, dando respiro strategico e forte valenza operativa alla *partnership* Italia-Libia. La mozione che ho firmato insieme a numerosi altri colleghi e che trova felice riscontro in altro analogo documento, chiede ora al Governo di dare seguito concreto a quella decisione, negoziando con la Libia, in tempi ragionevolmente brevi, i tre punti che ho indicato. Concludo, signor Presidente, ricordando che nel 2003 le intese italo-libiche furono realizzate dal Governo Berlusconi nello spirito di una lineare continuità con gli accordi di Roma del 13 dicembre 2000, firmati dal precedente Governo di centro-sinistra. Nel segno di una eguale continuità, come si addice alle grandi decisioni di politica estera, chiediamo ora al Senato, chiediamo ora al Senato, alla maggioranza e al Governo di dare attuazione alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio scorso. Proprio per questo, chiediamo al Senato un consenso largo, un consenso che avrebbe esclusivamente il significato di un atto di fiducia nel rilancio dei rapporti italo-libici e costituirebbe sicuramente un contributo significativo

soltanto confermare l'orientamento del Gruppo dell'Ulivo a sostegno delle ragioni di un voto di quest'Aula, la cui opportunità, che è stata egregiamente illustrata dal presidente Dini, nasce sicuramente da esigenze di carattere specifico che sono state richiamate nel corso della discussione, su cui tornerò molto rapidamente, ma anche da ragioni di carattere generale, di fondo. Noi stiamo attraversando una fase estremamente delicata della vita mondiale e lo stesso dibattito politico del nostro Paese è fortemente segnato, proprio in queste ore ed in questi giorni, da una discussione relativa a scelte cruciali di politica estera, nelle quali, indipendentemente dai punti di vista, vi è un dato che accomuna, credo, tutti i protagonisti di tale discussione, e cioè la necessità e l'esigenza di assegnare al nostro Paese un ruolo cruciale nella costruzione di un mondo che sia un mondo di pace. In questo quadro, il ruolo che spetta al nostro Paese viene dalla sua collocazione geografica, dall'essere cioè un Paese situato al centro del Mediterraneo;

In tale ambito, si colloca il lavoro che si è svolto e che si deve svolgere in maniera più intensa nel rapporto tra l'Italia e la Libia. Naturalmente ci sono anche ragioni più specifiche: vi è la necessità di consolidare questo rapporto per rendere più forte la lotta al terrorismo

clandestina. Altre ragioni molto specifiche riguardano gli interessi del nostro Paese e cioè la necessità di chiudere positivamente e di risolvere la questione che riguarda il rientro dei beni degli italiani ed il ristoro dei crediti per le attività economiche già svolte. così come si ricordava, nel quadro di un tormentato rapporto tra questi due Paesi, in tutto il dopoguerra la forza dell'Italia è stata quella di non avere mai smarrito un legame di amicizia e di

ed io mi auguro che aiuti quel Paese anche a superare i problemi ancora irrisolti sul terreno del rispetto dei diritti umani e dello sviluppo della democrazia.

come ha giustamente richiamato il presidente Dini, in quel comunicato congiunto del 1998 l'inizio di una più stringente azione di collaborazione

un gesto anche di umiltà e di disponibilità a chiudere la pagina di una brutta storia che, come giustamente si ricordava, condiziona ancora, con la sua memoria, le vicende dei rapporti fra i nostri due Paesi. Questo rapporto è poi andato avanti,

torna utile e necessario al nostro Paese. Si rende, cioè, ormai non più rinviabile la definizione,

che possa cancellare definitivamente dalla memoria quella brutta storia che segna il rapporto tra i nostri due Paesi.

delle valutazioni e delle analisi che per alcuni aspetti sono - ahimè, guai se così non fosse - anche articolate,

si creano condizioni e messaggi così forti e unitari, il Governo trovi più ragioni di incoraggiamento per andare avanti nella strada che ha già intrapreso, che il Sottosegretario ha qui egregiamente illustrato e che io credo possa rappresentare la linea alla quale ispirare l'azione dell'Italia nei prossimi mesi.

perché entrambe pongono alla nostra attenzione la necessità innanzitutto di dar seguito all'impegno del Governo del 23 febbraio del 2006 che - come è stato ricordato dai colleghi pone definitivamente fine al contenzioso fra il nostro Paese e la Libia e chiude un capitolo della nostra storia qual è stato quello del colonialismo. l'attenzione che l'Italia riserva a questo grande Paese del Mediterraneo, soprattutto di fronte agli avvenimenti dell'attualità, debba essere rafforzata anche dal nostro voto parlamentare. stati anni difficili in cui la Libia si era collocata nel contesto del Mediterraneo come elemento di rottura

credo, anche con le missioni del Presidente del Consiglio nel 1999 e poi con quelle di Berlusconi negli anni dal 2001 al 2006,

un'utile cerniera per l'intera Europa e per il mondo occidentale per poter parlare a quei Paesi che oggi nel Mediterraneo si trovano a guardare ad un'Europa che rischia di essere sempre più distante dai loro problemi. È con questo spirito che il nostro Gruppo voterà con convinzione la mozione del senatore Pisanu

La seduta è tolta